Dopo l'illustrazione delle mozioni, ciascun Gruppo avrà a disposizione venti minuti, comprensivi dei tempi della discussione e delle dichiarazioni di voto. Come preannunciato nella seduta antimeridiana di oggi, le votazioni avranno luogo non prima delle ore 18,15. Ha facoltà di parlare la senatrice Amati per illustrare la mozione n. 3. Il fatto che il 2008 sia l'anno del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ed anche l'anno del 60° anniversario della Costituzione repubblicana, ci impone, con ancora più forza, di operare affinché i diritti umani non restino solo una dichiarazione, ma si sostanzino nell'affermazione e promozione di una cultura e di una politica di cui il Senato deve farsi protagonista. Questo vuol dire rivolgere il nostro impegno alle molte centinaia di migliaia di persone condannate a morire di fame, sete, malattie, violenze, torture e guerre, vittime innocenti di armi micidiali. È questa cultura che vive nell'intervento che Benedetto XVI ha già fatto a Genova, indirizzando un appello contro le bombe a grappolo. Anche le istituzioni repubblicane debbono far sentire forte e chiara la loro voce. II Papa si è rivolto alla Conferenza internazionale di Dublino, ancora in corso, con l'invito che si potesse «rimediare agli errori del passato ed evitare che si ripetano in futuro», auspicando che la Conferenza potesse «produrre una Convenzione che interdica questi micidiali ordigni». Alla Conferenza, proprio sul tema della messa al bando delle bombe a grappolo, partecipano oltre cento Stati membri delle Nazioni Unite. Numerosi i temi nell'agenda della Conferenza che prevedono, oltre la messa al bando, anche che si stabilisca un quadro per l'assistenza ai sopravvissuti, che si fissi un programma di bonifica delle aree contaminate, e che si provveda alla distruzione delle riserve di queste armi. Tutta la comunità internazionale spinge per la soluzione di questo problema, che vede ancora molte industrie impegnate nella produzione di armi a grappolo e molti eserciti utilizzarle. Per quanto riguarda l'Italia, essa è uno dei 57 Paesi che ha in deposito tali ordigni e uno dei 32 Paesi che li producono. Le munizioni *cluster* sono armi di grandi dimensioni che si aprono a mezz'aria spargendo ad ampio raggio centinaia di submunizioni più piccole. Le submunizioni sono progettate in modo da esplodere al momento dell'impatto al suolo e questa è la differenza teorica con le mine antipersona, che sono progettate per essere attivate dal contatto con la vittima. Tuttavia, in molti casi le submunizioni non funzionano come previsto, restano inesplose sul terreno e quindi possono esplodere al minimo contatto diventando così di fatto mine antipersona. Il tasso di mancata esplosione dichiarato dalle case produttrici è del 5 per cento, ma in realtà i dati raccolti sul campo segnano indici molto più alti, fino al 20-25 per cento. Questo tasso è influenzato da fattori tecnici ed anche da condizioni ambientali, del terreno e dell'altezza da cui sono stati lanciati gli ordigni. Un esempio: nella seconda guerra del Golfo risulta siano state usate oltre 10.000 munizioni *cluster*, per un totale di circa 1.800.000 submunizioni. Se anche quelle inesplose fossero solo il 5 per cento, si tratterebbe comunque di 90.000 ordigni letali disseminati sul terreno. Per venire a un conflitto più recente, nel Sud del Libano risulterebbero 100.000 submunizioni inesplose. Le operazioni di bonifica risultano poi comunque complesse, sia per la difficoltà dell'identificazione, sia per l'oggettiva pericolosità. Possiamo ricordare le operazioni di bonifica condotte in Adriatico nel maggio 1999 per consentire il ripescaggio di decine di submunizioni rilasciate da aerei NATO dopo le missioni in Serbia e in Kosovo in manovre di emergenza. La nostra mozione, dunque, ha l'obiettivo di impegnare il Governo a che il nostro Paese, presente alla Conferenza internazionale di Dublino, assuma una posizione netta in favore della messa al bando delle *cluster bomb* e a sviluppare a tal fine un'iniziativa diplomatica per coinvolgere la comunità internazionale nell'adozione di uno strumento giuridicamente vincolante, che vieti senza ambiguità l'uso, la produzione, il trasferimento, la vendita e lo stoccaggio delle munizioni a grappolo.

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo e onorevoli colleghi, nel mondo, in questa fase storica di mutamenti epocali, continuano a verificarsi conflitti armati tra Stati, o ancor più interstatali, che coinvolgono soprattutto le popolazioni civili, già spesso piegate dal sottosviluppo e dal bisogno economico. Nonostante le precise indicazioni del diritto internazionale umanitario, espresse dal I e II Protocollo addizionale della Convenzione di Ginevra del 1949, per la protezione delle vittime nei conflitti armati internazionali e nei conflitti armati non internazionali, adottato a Ginevra l'8 giugno 1977 e ratificato in Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 762, all'interno di tali conflitti si verificano continue violazioni delle norme umanitarie, soprattutto per il proliferare dell'utilizzo delle *cluster bomb* o *cluster munition*, sistemi di arma progettati per rilasciare altre piccole bombe o submunizioni che possono essere utilizzate per una pluralità di funzioni (antiuomo a frammentazione, anticarro, antimateriali), ma comunque destinate a colpire a morte l'equipaggio, ad effetto combinato di frammentazione ed incendiario, per devastare intere aree, ove sempre, oltre all'obiettivo militare vi sono insediamenti della popolazione civile. La problematicità di tali armi sul piano umanitario, connessa con l'uso indiscriminato che a volte ne è stato fatto anche contro popolazioni civili, è accresciuta dalla loro relativa inaffidabilità. In effetti, una percentuale variabile delle munizioni lanciate non esplode al momento di colpire l'obiettivo e rimane sul terreno, trasformandosi in pericolosi residuati bellici esplosivi, comunemente chiamati dagli esperti *explosive remnant of war* (ERW), suscettibili di causare vittime anche nei periodi post-bellici. Una volta sul terreno, basta un nulla per farle esplodere, causando morti, mutilazioni e sofferenze a popolazioni civili, militari, forze di pace, sminatori ed in particolare a bambini, attratti dalla forma e dai colori vivaci di tali ordigni. Incalcolabili sono le sofferenze e le perdite di vite umane causate dall'uso di munizioni a grappolo, che uccidono o mutilano civili innocenti e inermi, soprattutto bambini, ostacolano lo sviluppo economico e la ricostruzione, ritardano o impediscono il ritorno dei profughi e degli sfollati e provocano altre gravi conseguenze umanitarie che possono persistere per molti anni dopo l'uso di siffatti ordigni. Ingenti danni, soprattutto ai civili, sono stati provocati negli ultimi tempi in particolare in Libano, Iraq, Kosovo, Laos, Afghanistan, Angola. Nel rapporto del 2008 di Amnesty International, presentato in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, viene sottolineato come la violazione dei diritti umani rimane un fenomeno costante in gran parte del pianeta. Il forte impegno della comunità internazionale, realizzato attraverso le Nazioni Unite e le organizzazioni regionali, in particolare l'Unione Europea, per costruire un sistema di sicurezza e pace internazionale attraverso le missioni di *peace keeping* e di *peace building* rischia di essere indebolito dagli effetti devastanti delle *cluster munition*, che contrastano con i processi in atto per la protezione ed il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei Paesi lacerati dai conflitti. Già da tempo le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per l'impatto umanitario delle *cluster bomb*, i loro effetti indiscriminati e l'imprevedibile funzionamento. In particolare, è da citare la posizione espressa nella riunione dei rappresentanti ONU del 17 settembre 2007, in cui le Nazioni Unite hanno invitato gli Stati membri ad affrontare immediatamente gli effetti devastanti delle munizioni a grappolo sul piano umanitario, dei diritti umani e dello sviluppo. L'Italia è stata sempre impegnata a livello internazionale per pervenire alla messa al bando di queste armi definite disumane, partecipando sia alla Convenzione su «Certe Armi Convenzionali (CCW)» di Ginevra del 1980, sia al "Processo di Oslo" avviato nel 2007 e sviluppatosi attraverso le Conferenze di Oslo, Lima, Vienna, Wellington e Dublino, aperta il 19 maggio 2008 ed ultima tappa del processo per definire un trattato internazionale che preveda il divieto dell'uso, della produzione, del trasferimento e dello stoccaggio delle munizioni a grappolo. Forti sono le aspettative al riguardo da parte degli organismi e degli Stati finora impegnati su tale fronte e si è pronunciato al riguardo più volte anche il Parlamento europeo. Il giorno precedente l'apertura dei lavori della Conferenza diplomatica di Dublino un significativo messaggio agli Stati partecipanti è arrivato anche da Papa Benedetto XVI, che ha auspicato la definizione di una Convenzione per interdire tali armi micidiali. E' di queste ore la notizia che anche la Gran Bretagna è disponibile a dare il proprio contributo nella Conferenza ed a smantellare l'intero arsenale di bombe a grappolo. I lavori di Dublino assumono ancora maggiore importanza per la pace e la sicurezza internazionale anche alla luce delle recenti minacce mediatiche lanciate dal *network* terroristico di Al Qaeda di utilizzare armi di distruzioni di massa nei confronti delle popolazioni civili dell'Occidente. L'Italia, unitamente alle Nazioni Unite ed all'Unione Europea, per l'impegno internazionale profuso negli anni a favore dei diritti umani, ha il dovere di svolgere un ruolo propulsivo fondamentale nel corso della Conferenza di Dublino di convincimento e coinvolgimento degli altri Paesi presenti, per la definizione di un trattato internazionale quale valido strumento giuridicamente vincolante per vietare l'uso, la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio delle munizioni a grappolo, stabilire un quadro di cooperazione di assistenza, di riabilitazione per i sopravvissuti e le loro comunità,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono centinaia i diplomatici e le organizzazioni non governative provenienti da tutto il mondo attualmente impegnati a Dublino nell'elaborazione di una bozza definitiva per mettere finalmente al bando gli orribili ordigni che portano il nome di *cluster bombs*, ossia bombe a grappolo. Tengo a sottolineare che la Conferenza internazionale di Dublino ha ricevuta la benedizione, il sostegno, la preghiera del sommo Pontefice Benedetto XVI, il quale ha espresso l'auspicio di poter presto giungere ad un accordo internazionale su questi terribili ordigni. La Conferenza di Dublino dovrebbe, dunque, rappresentare l'ultima e cruciale tappa di un lungo e travagliato processo che cominciò ad Oslo nel 2007 e che nel febbraio 2008 ha portato 81 Paesi, tra cui l'Italia, alla Dichiarazione di Wellington. La cosiddetta campagna italiana contro le mine considera questa Dichiarazione una bozza soddisfacente per il testo del trattato che - spero - verrà a breve negoziato e concordato a Dublino. Se, come si attende, la Conferenza giungerà alla redazione di una bozza definitiva, tale documento costituirà il più importante trattato per il disarmo dalla Convenzione di Ottawa,

che alla Conferenza di Dublino non partecipano alcuni tra i maggiori produttori di *cluster bombs* come gli Stati Uniti, la Russia, l'Israele, la Cina ed il Pakistan, i quali non firmarono neanche la Dichiarazione di Wellington. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti sappiamo che le bombe a grappolo sono armi pericolosissime, di grandi dimensioni, sganciate da aerei o esplose da sistemi di artiglieria, da lanciarazzi e lanciamissili,

I modelli più comuni sono stati concepiti in funzione antiuomo e antiblindatura. Altri tipi di bomba a grappolo vengono utilizzati per distruggere infrastrutture militari o civili, linee di trasmissione elettrica, disperdere armi chimiche o biologiche e disseminare il terreno di mine antipersona. Questi ordigni hanno una capacità di dispersione in un'area molto vasta e la durata nel tempo del loro effetto è letale. letale. Inesplose possono rimanere attive per molti anni contaminando il terreno al pari delle mine antiuomo. Si stima che queste bombe, utilizzate negli ultimi anni in tutto il mondo, abbiano causato centinaia di migliaia di morti. di morti. Signor Presidente, è vero che l'Italia si annovera tra i Paesi più attivi per la messa al bando di queste mine antiuomo, tuttavia si annovera anche tra quei Paesi che hanno nei propri arsenali munizioni *cluster*. Mi preme, inoltre, ricordare che l'Italia ha partecipato e partecipa tuttora a missioni internazionali nelle quali è stato fatto uso da parte di forze alleate di tali armamenti. L'Italia, e ciò mi rincresce ancor di più, risulta anche fra i Paesi produttori; tutti ricordiamo la sconvolgente inchiesta condotta da Rainews 24, che smascherò un'azienda italiana che esportava componenti di *cl**uster*. Signor Presidente, onorevoli colleghi,

non solo per richiedere con fermezza la messa al bando di queste armi, ma anche di mettere in atto una sorta di operazione convincimento al fine di spingere anche gli altri Paesi a vietare una volta per tutte la produzione e l'utilizzo di questi terribili ordigni. Mi preme sottolineare che apprezzo molto l'impegno comune di tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione che all'unisono chiedono una svolta. Ho firmato con convinzione la mozione anche perché da anni sono impegnato in tal senso. Ho sottoscritto già nel 2006 un disegno di legge, ripresentato

esplosivi (allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980). Questo nuovo Protocollo intende ridurre il più possibile i pericoli e gli effetti dei residuati bellici esplosivi per le popolazioni civili. Esso prevede, per gli Stati sul cui territorio si trovano residuati bellici esplosivi, l'obbligo di bonifica del territorio e l'obbligo di contribuire alla bonifica fornendo un'assistenza tecnica e finanziaria. Stabilisce inoltre l'obbligo di registrare e archiviare le informazioni sulle munizioni esplosive impiegate e di scambiare informazioni allo scopo di facilitare la bonifica. Il Protocollo, che l'Italia dovrebbe ancora ratificare, definisce infine una serie di misure per avvertire le popolazioni civili del potenziale di rischio rappresentato dai residuati bellici esplosivi. Ci tengo a precisare che il Protocollo è perfettamente compatibile con il nostro ordinamento giuridico. Onorevole Presidente, cari colleghi, sia le considerazioni umanitarie, sia l'attuale assenza nel diritto umanitario internazionale di regole pertinenti depongono a favore di una sua ratifica. Approfitto, dunque, di questa occasione non solo per annunciare il voto favorevole dei membri del Gruppo UDC, SVP e Autonomie alle mozioni in discussione quest'oggi, ma anche per chiedere un celere esame del disegno di legge da me presentato perché certo del vostro sostegno. Sarei lieto, inoltre, se i colleghi senatori indipendentemente dalla loro appartenenza ad un Gruppo parlamentare seguissero il nostro invito a firmare il disegno di legge per la ratifica del Protocollo del 2003. Ringrazio i colleghi per l'attenzione.

Signor Presidente, onorevoli senatori, è questa la prima volta che ho l'onore di parlare in quest'Aula del Senato e lo faccio a sostegno della mozione n. 3, presentata dalla senatrice Pinotti e da altri colleghi del Partito Democratico. È una mozione che chiede al Governo di assumere una forte e incisiva azione per la messa al bando delle *cluster bomb*. Stiamo parlando di munizioni particolari, che si differenziano dalle altre in quanto non sono dirette contro un singolo bersaglio militare, ma determinano la dispersione e la distribuzione su ampie superfici di terreno di centinaia di ordigni esplosivi, di limitate dimensioni ma di alta capacità distruttiva e di offesa. La guerra è l'evento più tragico delle relazioni umane; un evento che porta con sé distruzioni, sofferenze e morte; tutti lo sappiamo. Le controversie internazionali o interne ai Paesi dovrebbero essere superate ricorrendo al confronto pacifico delle posizioni, al dialogo, alla ricerca di punti di possibile convergenza. Anche di questo tutti siamo consapevoli, ma tutti sappiamo anche che purtroppo non sempre è così. Oggi, all'inizio del terzo millennio, la vita del mondo contemporaneo è segnata tristemente da un numero elevato di conflitti. In questa realtà di per sé drammatica, nella quale invero l'Italia cerca di dare un contributo alla risoluzione delle crisi con l'azione della politica e con l'impegno dei propri contingenti militari, esistono purtroppo esistono purtroppo circostanze nelle quali vengono impiegati strumenti che mirano a colpire indiscriminatamente, senza alcuna distinzione tra combattenti e non combattenti. strumenti che non hanno alcun riguardo nei confronti dei civili inermi e che quindi, proprio perché civili ed inermi, non dovrebbero essere coinvolti nelle guerre. Vengono utilizzati ordigni che non si limitano a colpire al momento dell'impiego, ma che continuano a produrre i loro tragici effetti sulle popolazioni civili spesso molto tempo dopo la fine del conflitto stesso, quando le popolazioni che hanno già subito pesantemente le sofferenze della guerra credono e sperano di aver finalmente riconquistato la pace. È questo il caso delle *cluster bomb*. Onorevoli senatori, non c'è alcuna logica militare nel loro impiego perché sono ordigni che non hanno capacità risolutiva; nel loro impiego c'è solo il completo spregio di ogni considerazione di carattere umanitario. Il fatto che le vittime più numerose di queste munizioni siano le persone più deboli ed indifese ed i bambini - e chi vi parla, purtroppo, ha potuto rendersi direttamente conto di questa realtà sottolinea ancora di più, se ce ne fosse bisogno, l'assurdità dell'impiego di questi ordigni. Non è solo il nostro umano sentire che ci porta a condannare le *cluster bomb*, sono le Convenzioni di Ginevra che ci ricordano l'assoluto divieto degli attacchi militari indiscriminati, che ci ricordano ancora il divieto degli attacchi con metodi che non hanno un obiettivo militare determinato. È, quindi, nostro dovere - così almeno io percepisco questa discussione - operare perché venga posta fine a questa violenza indiscriminata, assurda e ingiustificabile. Credo che sia nostro compito, onorevoli senatori, percorrere anche in questa circostanza la via della civiltà che l'Italia ha già seguito numerose volte; percorrere quella stessa via della civiltà che indusse i nostri predecessori nel Parlamento nazionale nel 1997 a bandire le mine antipersona. Onorevoli senatori, richiamando questi principi di civiltà e di umanità, formulo quindi la speranza che vogliate sostenere la mozione di bando delle munizioni a grappolo, dalla senatrice Pinotti e da altri senatori, senza subordinare la decisione agli orientamenti di altri soggetti o di organismi esterni a quest'Aula ed all'Italia, anzi cercando di convincere coloro che, su questo argomento, non hanno la nostra al Governo italiano un forte mandato per operare ancora una volta efficacemente in un contesto internazionale, combattendo e possibilmente vincendo un'altra battaglia di civiltà.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, premetto innanzitutto che quando si parla di armi, di strumenti che colpiscono indiscriminatamente anche le popolazioni civili, per quella che è la mia, la nostra cultura, non si può non inorridire. Bene ha fatto il Santo Padre a porre nei giorni scorsi al centro dell'attenzione mondiale il problema della messa al bando di questo tipo di armi, appunto delle bombe a grappolo. Non voglio qui scendere nel dettaglio tecnico di utilizzo di queste bombe, che sono di vario tipo e vengono utilizzate in differenti condizioni dal punto di vista strategico, e tale utilizzo chiaramente diverso determina delle ricadute diverse sulla popolazione civile; voglio innanzitutto, prima di continuare il mio intervento, sottolineare l'assoluta contrarietà della Lega Nord all'utilizzo di questo tipo di armi. però, tenere presente anche gli accordi internazionali e i rapporti con i Paesi alleati dell'Italia: nei confronti dell'ipotesi di un bando completo ed indistinto, purtroppo, non c'è consenso unanime nella comunità internazionale. Vediamo ad esempio la Federazione russa, che ha deciso di disertare la Conferenza di Dublino, così come ha deciso di fare la Repubblica popolare cinese, ma sono emerse anche delle differenze all'interno dell'Alleanza atlantica e addirittura all'interno dei singoli Governi di Stati membri,

privarsi delle *cluster bomb*: la Difesa britannica, ad esempio, che utilizza bombe a grappolo capaci di

ritorsioni che potrebbero avere delle conseguenze, per esempio le limitazioni delle esercitazioni interalleate o delle stesse azioni combinate

Non possiamo escludere o non possiamo assolutamente rischiare, per esempio, che nella provincia di Farah, qualora i nostri soldati si ritrovino in difficoltà, gli americani rinuncino ad intervenire a supporto delle nostre truppe magari come atto di ritorsione per un nostro atteggiamento estremamente intransigente a Dublino. Questo non vuol dire una posizione arrendevole nei confronti di Washington, assolutamente; ma bisogna dimostrare realismo e bisogna cercare di tutelare la causa del diritto bellico e comunitario senza sfidare il buonsenso. Circoscrivere il bando totale alle munizioni a grappolo che provocano sofferenze inaccettabili alle popolazioni civili, va esattamente in questa direzione

Signora Presidente, colleghi senatori, dopo le parole della senatrice Amati e soprattutto dopo l'intervento così chiaro, profondo e forte

che l'azione per la pace e per i diritti umani non è solo quella che si svolge nell'alternativa tra pace e guerra, ma

il Corano prescrive: non distruggerai i raccolti e non avvelenerai i pozzi dei tuoi nemici; ciò a indicare il limite che la legge e la coscienza morale devono

del principio dellatutela dei diritti e della sicurezza umana come elemento caratterizzante del comportamento dei Paesi civili anche dentro le fasi di conflitto sono elementi essenziali. Noi siamo alla vigilia della difficile discussione sulla questione delle nostre missioni internazionali e delle regole di ingaggio, ma in questa discussione il problema della sicurezza umana e del rapporto con le popolazioni civili, il problema cioè di un'azione e di una presenza nei conflitti orientate alla protezione delle popolazioni civili, che non consideri indifferente la propria azione (ricordo che oggi nei conflitti moderni la maggioranza delle vittime non sono militari ma cittadini

dentro i conflitti discutiamo non solo nel nostro Paese ma nell'insieme del sistema di alleanze di cui noi siamo parte. Vorrei concludere con una considerazione politica. Oggi su questo tema

Ringrazio il senatore Mura per la chiarezza con cui ha posto tale questione al di fuori di qualsiasi infingimento. Voi in sostanza ci proponete una mozione che dice: siamo disposti a prendere una posizione, a condizione che

della difesa e degli esteri oltre che ascoltare, come è giusto, necessario e doveroso, i Capi di Stato maggiore, ascoltassero anche i soldati e gli ufficiali italiani che in Libano sono impegnati ad insegnare ai bambini come evitare i pericoli che minacciano la loro vita, forse oggi ci proporrebbero una posizione

Presidente, ho ascoltato gli interventi precedenti, alcuni dei quali, come quello del mio amico generale Del Vecchio, mi risparmiano di entrare nel merito tecnico della questione,

Hanno dunque un significato operativo, ma un significato operativo lo avevano anche le mine: non è che fossero un'arma decaduta come importanza. Anche le mine avevano un loro significato operativo, anzi direi che ne avevano uno anche maggiore di questo, che è un particolare tipo di sistema d'arma, tipo di sistema d'arma, che però rischia di diventare, anzi in realtà diventa, assolutamente nefasto nei confronti della popolazione civile che vive nelle aree soggette a simili interventi durante le operazioni belliche. Tutti noi abbiamo visto quello che ci hanno mostrato i nostri militari impegnati in Libano nell'opera di bonifica, ma sono 30 i Paesi che stanno soffrendo per questa realtà.

debbo dire che questi sistemi di distribuzione di ordigni, a volte, sono anche volutamente indirizzati a far sì che non esplodano immediatamente, ma che esplodano a tempo

sono due mozioni che praticamente dicono la stessa cosa e questa convergenza mi fa doppiamente piacere.

una soluzione giuridicamente vincolante, condivisa in sede internazionale, che proibisca la produzione e naturalmente il conseguente impiego

Il problema riguarda apparentemente poche parole, forse una decina, che differenziano la mozione della maggioranza rispetto a quel che vede come prima firmataria la senatrice Pinotti. Non devo fare la storia, che è già stata ricordata abbondantemente, vorrei solo dire che la posizione finora assunta dal Governo italiano, in assoluta continuità con il Governo precedente, fa riferimento ad un atto parlamentare di grande significato, che è stato compiuto nella scorsa legislatura, quando la Commissione affari esteri della Camera ha adottato all'unanimità - ci tengo a sottolinearlo - la risoluzione presentata dall'onorevole Siniscalchi. Il problema è molto semplice. Oggi i sostenitori del "Processo di Oslo" sono circa 119; mancano Stati Uniti, Russia, Cina, India, Pakistan, Israele e Brasile. Non è purtroppo la prima volta nel campo dei problemi riguardanti gli armamenti che i grandi Paesi mancano all'appello rispetto alla grande comunità internazionale.

di una stretta concertazione con i *partner* nelle operazioni di pace delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza Atlantica, anche in relazione alle esigenze di integrazione reciproca,

che, in fondo, l'atto parlamentare avrebbe un maggiore significato se vi fosse unanimità sulle mozioni, vorrei dire con grande chiarezza che il tema è tra la volontà assolutamente decisa del Governo italiano e la realtà nella quale noi operiamo. Noi possiamo benissimo far finta di non sapere di essere impegnati in operazioni di pace sotto egide multilaterali. Molte delle operazioni di pace attualmente in corso sono ampiamente condivise da maggioranza ed opposizione. Non possiamo, però, fare finta di non sapere che insieme a noi vi sono forze armate alleate facenti capo a Paesi che sulle *cluster* *bomb* nutrono - purtroppo - un'opinione diversa dalle nostre.

a batterci per l'eliminazione di questo tipo di arma. Voglio ricordare anche qui che, con assoluta continuità nelle varie formule governative, la campagna contro le mine antiuomo vide l'Italia fra i primi Paesi a raggiungere l'obiettivo di distruzione dei propri magazzini. Voglio anche

assolutamente lo spirito della mozione presentata a prima firmataria dalla senatrice Pinotti, inserisce un elemento di cautela ed attenzione che risponde doverosamente e obiettivamente ad esigenze che tutti noi conosciamo. Peraltro, il Governo è costretto a dire che approva, sottoscrive ed accetta la mozione di maggioranza, e auspica che i colleghi dell'opposizione si sentano soddisfatti dalla risposta data dal Governo e che si possa trovare assieme una soluzione

GIAMBRONE *(IdV)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori vorrei esprimere pochi e semplici concetti per motivare il nostro voto favorevole alla mozione, avente come prima firmataria la senatrice Pinotti, di cui oggi discutiamo in quest'Aula. Innanzitutto, il Gruppo dell'Italia dei Valori intende porre l'accento sull'importanza del raggiungimento degli accordi internazionali che perseguono efficacemente gli obiettivi che si prefiggono. È questo, infatti, il caso della Conferenza in corso a Dublino riguardante le *cluster munition*, ma è anche il caso delle cosiddette Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e, in particolare, della IV Convenzione sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra. Queste Convenzioni, infatti, a pochi anni dalla fine della seconda guerra mondiale hanno sostituito tutto il corpo giuridico preesistente in materia. Occorre ricordare, colleghi, che quasi 100 anni prima delle Convenzioni del 1949, nel 1859, a seguito degli orrori generati da un'epica battaglia - quella di Solferino - combattuta tra l'esercito austriaco e quello franco-sardo, alla quale presero parte più di 200.000 soldati, si diede vita, grazie ad una lunga serie di trattati, ad un corpo giuridico di diritto internazionale, che poi è andato sotto il nome di Diritto di Ginevra, o Diritto delle vittime di guerra e internazionale umanitario. Tralasciando i pur interessanti passaggi storici e prettamente relativi al diritto internazionale, il Gruppo dell'Italia dei Valori vuole, in questa dichiarazione, richiamare l'attenzione dei colleghi parlamentari sull'importanza del testo in esame, per la cui presentazione vorrei ringraziare la collega Pinotti che ha il merito di averci costretto ad occuparci di un avvenimento che si svolge in questi giorni ma del quale i media spesso non parlano. Vorrei, dunque, richiamare l'attenzione dell'Aula sul testo in esame, non tanto per il suo meritevole contenuto ma in quanto per il più generale sforzo di impegnare il governo nazionale al raggiungimento, nella sede preposta di Dublino, di un accordo per l'effettiva messa al bando delle bombe a grappolo. Dico "effettiva", colleghi, perché, come molti di voi sapranno, troppe volte le conferenze internazionali si concludono con accordi al ribasso. Non solo; oltre a questo è necessario, come nel caso dell'Italia, che i Parlamenti ratifichino tali accordi, presi quasi sempre almeno una decina di anni prima. È questo un punto su cui l'Italia dei Valori vuole che il Governo italiano faccia valere la sua forza e sappia far notare la differenza sostanziale tra gli Stati circa gli impegni presi, evitando accordi al ribasso ed essendo da traino per i Paesi, purtroppo molto importanti nello scacchiere internazionale, che ancora oggi non siedono a Dublino. È molto importante che il Governo vada a sostenere una posizione chiara, senza ambiguità alcuna, in favore della messa al bando delle cosiddette bombe a grappolo, del loro uso, produzione, trasferimento, vendita e stoccaggio. Inoltre, il nostro Paese dal 1997 ha adottato la legge n. 374, che prevede la messa al bando delle mine antipersona. Credo che il contenuto della legge in questione - mi rivolgo alla collega Pinotti - non solo «appaia riferibile», come riportato nel testo della mozione, ma sia completamente assimilabile, ovviamente per ciò che concerne le conseguenze dell'utilizzo. Il problema consiste però non solo nel migliorare la normazione interna a tutti i livelli (si potrebbe quindi anche migliorare il testo della legge n. nel portare gli altri Stati a sostenere a livello di trattati internazionali, come quello a cui si dovrebbe arrivare a Dublino, le tesi contenute nella mozione della collega Pinotti. come credo risulti anche a voi e come leggo nella premessa della mozione a firma della senatrice Pinotti, che proprio in Libano, dove i nostri soldati sono ormai da tempo impegnati in una missione internazionale tra le più importanti e delicate per le relazioni internazionali del nostro Paese (missione che peraltro guidiamo dal 2007), siano sparsi, secondo stime di diverse organizzazioni internazionali tra le quali anche l'ONU, almeno 100.000 ordigni inesplosi. Bene, colleghi! Tralasciando (ma non perché non importante, anzi al contrario) il fatto che i nostri militari hanno tra i loro compiti precipui proprio la bonifica del territorio (quindi dovrebbero essere quanto meno preparati a farlo), il problema dalle proporzioni enormi che comporta l'utilizzo di queste bombe è la pericolosità delle stesse per la popolazione civile. Secondo un rapporto di *Handicap International*, nel mondo le vittime delle bombe a grappolo sono per il 98 per cento civili e, sparse su tutto il pianeta, dovrebbero esserci qualche centinaio di milioni, ripeto colleghi, qualche centinaio di milioni di esemplari di questo genere di munizioni. Soltanto gli Stati Uniti, peraltro neppure presenti ai negoziati di Wellington in Nuova Zelanda, pare posseggano tra i 700 e gli 800 milioni dì questi ordigni, che immagino abbiano interesse a smaltire, con tutto il loro carico di morte, prima della riuscita di questa importante Conferenza internazionale. Mi risulta da fonti, tra le più importanti, dell'associazionismo a fini umanitari che ci sia addirittura chi a Dublino vuole sostenere la moratoria solo per gli armamenti di questa tipologia di vecchia concezione, come se le bombe a grappolo di nuova generazione possano esser ritenute intelligenti intelligenti tanto da capire che non devono scoppiare in mano ad un bambino che si china per coglierle o di colui che ci mette il piede sopra mentre gioca a pallone. Vedete colleghi, avendo poco più di quarant'anni e, soprattutto, avendo avuto la fortuna di non vivere le

nuova generazione, quindi più o meno sicure o, ancora, tra bombe più o meno problematiche per le loro conseguenze. Occorre, come ho anticipato nel prologo del mio intervento, che in seno alla Conferenza di Dublino il Governo italiano sposi la tesi della definitiva cessazione della produzione, uso, sviluppo e quant'altro di queste bombe, all'interno di un Trattato vincolante, quale quello che scaturirà dagli incontri di Dublino di questi giorni. Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori alla mozione n. 3 a firma della senatrice Pinotti. *(Applausi

Presidente, onorevoli colleghi, sappiamo tutti che nel primo protocollo aggiuntivo delle Convenzioni di Ginevra del 1949 alcune disposizioni vietano, tra l'altro, gli attacchi militari indiscriminati a danno delle popolazioni civili e quelli realizzati con metodi o mezzi di combattimento che non abbiano un obiettivo militare determinato. In questa ampia definizione è ovvio che vi possano rientrare numerosi sistemi d'arma prodotti negli ultimi sessant'anni, dagli ordigni nucleari alle stesse bombe a grappolo, meglio definite come *cluster bomb*. Bene ha fatto il Santo Padre nei giorni scorsi ad intervenire contro l'uso di questo tipo di armamento, anche perché grazie alla sua autorevolezza ha portato la comunità internazionale ad affrontare la questione della sua messa al bando. È evidente a tutti che la loro capacità di colpire obiettivi di area, piuttosto che precisi bersagli, accresce il rischio di colpire anche popolazioni civili e di causare effetti indiscriminati ed incompatibili con il diritto umanitario. Le *cluster bomb*, per le loro caratteristiche intrinseche, rendono difficile ed impossibile rispettare le norme del diritto umanitario. L'esempio più recente degli effetti negativi dell'utilizzo di queste bombe si è verificato in Libano, dove - è vero - sono rimasti sul terreno circa 100.000 ordigni inesplosi, che potrebbero determinare un effetto devastante tra la popolazione civile. La Lega Nord ribadisce il concetto della contrarietà all'utilizzo di queste bombe ed invita il Governo a tenere un atteggiamento deciso nei confronti della comunità internazionale per arrivare alla definitiva messa al bando delle bombe a grappolo. Purtroppo, però, va precisato ed ammesso che, rispetto all'ipotesi di un bando completo ed indistinto, non vi è un consenso unanime nella comunità internazionale. Tant'è vero che la Federazione Russa, in occasione della Conferenza di Dublino, che si prefiggeva come obiettivo il compito esplicito di pervenire all'adozione di «uno strumento giuridicamente vincolante che vieti senza ambiguità, l'uso, la produzione, il trasferimento, la vendita e lo stoccaggio delle munizioni a grappolo», ha disertato l'assemblea, così com'è stato fatto anche dalla Repubblica Popolare Cinese. Divisioni sono affiorate anche all'interno dell'Alleanza Atlantica e persino all'interno di alcuni dei Governi dei suoi principali Stati membri e, come ha già ricordato il mio collega di partito, senatore Mura, ribadisco che, in relazione agli impieghi delle stesse contro aeroporti e strade, alcuni Paesi non sono d'accordo a privarsi delle *cluster bomb*. Come è stato già citato, la difesa britannica, ad esempio, utilizza queste tipologie di bombe a grappolo, capaci di autodisinnescarsi se non esplodono al contatto. che gli stessi Stati Uniti hanno una posizione diversificata rispetto ad un bando totale. Tuttavia, visto che già dall'inizio di questa legislatura si è parlato di instaurare un clima di distensione politica, vorremmo suggerire all'opposizione di modificare l'impegno contenuto nella parte dispositiva della mozione Pinotti di prendere in considerazione l'eventualità di votare la mozione proposta dalla maggioranza che, raccogliendo il suggerimento del Governo, chiede che venga assunta nella Conferenza di Dublino, sulla base di una stretta concertazione con i *partner* nelle operazioni di pace delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza Atlantica, anche in relazione alle esigenze di integrazione reciproca, una decisa posizione a favore della messa al bando della *cluster bomb*. In mancanza di distinzioni adeguate, ritengo che la Conferenza di Dublino potrebbe invece partorire un accordo nocivo alla stessa tenuta dell'Alleanza Atlantica. È per queste ragioni che il Gruppo della Lega Nord Padania voterà

non si eserciteranno più nell'arte della guerra». La citazione scolpita sul monumento di fronte al Palazzo di Vetro si Isaia continua e prefigura uno scenario, ovviamente collocato nel mondo che verrà, dopo la fine della storia, in cui tutti i popoli si raduneranno attorno al Signore e sarà lui a giudicare i torti e le ragioni e tutti accetteranno questa sentenza e la guerra non avrà più quindi ragione d'essere. Ebbene, questo ideale, questa visione religiosa escatologica ha ispirato nel corso della storia un impegno fattivo contro la guerra. Il principale, più costruttivo impegno per la costruzione della pace, per la cancellazione della guerra dalla storia dell'uomo è quello della crescita del diritto, del diritto tra le genti, il diritto internazionale del quale il Palazzo di Vetro (pur così fragile come è il vetro

Ebbene, nella storia del diritto internazionale uno dei rami che hanno cercato di svilupparsi, di crescere, di diventare sempre più forti è stato il cosiddetto *ius in bello*, vale a dire il diritto della guerra e cioè il tentativo di limitare, attraverso norme, quella che è la più grande e clamorosa trasgressione della convivenza umana, che è l'esplosione della guerra. Perfino la guerra può, a certe condizioni e in certe circostanze, essere sottoposta alla signoria del diritto e comunque lo sforzo di sottoporre la guerra alla signoria del diritto non può mai venir meno,

un profilo tecnico l'utilizzo indiscriminato di queste armi. Armi che colpiscono uno dei princìpi e dei cardini dello *ius in bello* e cioè che non si debba mai fare uso di violenza indiscriminata contro le popolazioni civili, per di più con incerta connessione con precisi obiettivi di carattere militare. Pochi ordigni come le bombe a grappolo, le *cluster bomb* sono così patentemente e palesemente in violazione di questo principio fondamentale del diritto internazionale. Credo allora che sia un passaggio importante, quello che si sta verificando in questo momento nell'Aula del Senato. La maggioranza e l'opposizione, con testi diversi ma convergenti

ma sarebbe incomprensibile e impensabile che l'Italia assumesse una posizione che non fosse questa, di assoluta chiarezza. al sottosegretario Mantica, che sa quanto io apprezzi e stimi il suo lavoro e il suo impegno per rappresentare l'Italia nel mondo su una posizione certamente favorevole alla pace e alla costruzione della pace nel mondo, che c'è nel testo della mozione proposta dalla maggioranza un passaggio, un inciso che noi non ci sentiamo di condividere.

perfino scontato nel suo significato immediato. E il significato immediato è che noi non facciamo venire meno la solidarietà e la concertazione con le forze con le quali siamo alleati in tanti teatri di *peacekeeping*, a livello internazionale. È evidente che né questa mozione, né altri strumenti parlamentari possono e intendono in alcun modo mettere in discussione la nostra collocazione internazionale, il sistema di alleanze delle quali l'Italia fa parte, che si è andato rafforzando

cioè come se quell'inciso volesse attenuare il significato, la forza, la convinzione con cui l'Italia deve invece andare a quel negoziato. E tanto più questa amicizia, questa cordialità di rapporti con i nostri alleati è fuori discussione, tanto più deve essere invece netta la nostra posizione all'interno del negoziato di Dublino. Noi chiediamo quindi uno sforzo ulteriore alla alla maggioranza e al Governo affinché venga superata questa formulazione, che riteniamo debole. Quell'inciso finisce per indebolire il significato complessivo di nettezza del segnale politico che il Parlamento deve mandare al Governo. Chiediamo questo ultimo sforzo, nello spirito di convergenza che il Sottosegretario ha auspicato e che certamente ci trova molto sensibili.

Signora Presidente, colleghe e colleghi, caro Sottosegretario, il tema affrontato dalle due mozioni oggi discusse in quest'Aula testimonia la forte e chiara presa di coscienza da parte del Parlamento e del e del Governo italiano di un gravissimo problema, a cui la comunità internazionale ha da tempo dedicato energie ed impegno. Il Governo ed il Parlamento condannano severamente sotto l'aspetto etico e morale l'uso delle cosiddette bombe a grappolo. Su questo non ci piove: siamo assolutamente convinti, determinati

nella concertazione europea, nella condizione atlantica, dove noi orgogliosamente siamo da sempre presenti, oppure tutti questi distinguo non fanno altro che portare a opportunità

che proibisca la produzione e l'impiego delle *cluster bomb* rappresenta infatti un passo fondamentale nella direzione di una politica di disarmo a livello globale, globale, i cui primi frutti furono rappresentati dai contenuti della Convenzione di Ottawa del 1999, che ha proibito la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo delle mine antiuomo. Desidero quindi rivolgere un plauso particolare alla senatrice Pinotti, che nella scorsa legislatura, come giustamente il sottosegretario Mantica ha già sottolineato, quale Presidente della Commissione difesa della Camera dei deputati presentò in Commissione una risoluzione che, ricordo, fu approvata con un largo voto *bipartisan*. Quindi, noi votammo l'inibizione dell'uso delle *cluster bomb* da parte delle nostre Forze armate impegnate nelle missioni internazionali, nonché la promozione di una decisa azione diplomatica per vietarne la produzione, lo stoccaggio, il trasferimento e, soprattutto, l'uso. Il mio apprezzamento, se mi permettete, va anche ai colleghi dell'opposizione. A tale proposito ringrazio i senatori Del Vecchio, Marcenaro e gli altri che hanno preso la parola prima di me,

Come altri colleghi che mi hanno preceduto hanno già avuto occasione di ricordare, a Dublino è in corso la Conferenza per la messa al bando delle *cluster bomb* alla quale anche il nostro Sommo Pontefice, Benedetto XVI, ha dato la propria benedizione. Noi non solo ne teniamo conto, ma la consideriamo una angolazione fondamentale. Proprio la gravità delle tematiche connesse all'utilizzo di queste munizioni mi ha spinto, unitamente a tanti altri colleghi, che ringrazio per la sensibilità dimostrata,

sono solo le organizzazioni non governative impegnate nei diversi teatri di guerra a chiederlo a gran voce: ricordo che la comunità internazionale la comunità internazionale tutta ritiene ormai l'utilizzo di queste munizioni incompatibile con gli stessi princìpi generali del diritto internazionale. Bene ha fatto la senatrice Contini a ricordare le incalcolabili sofferenze, le perdite di vite umane causate da queste micidiali munizioni che uccidono o mutilano civili innocenti ed inermi e soprattutto - ahimè - i bambini, che ostacolano lo sviluppo economico e la ricostruzione, ritardano o impediscono il ritorno dei profughi e degli sfollati e provocano altri gravi conseguenze umanitarie che possono persistere per molti anni dopo l'uso di siffatti ordigni. Grazie, senatrice Contini. La mozione di cui sono firmatario correttamente riconduce l'impegno verso la messa al bando delle munizioni *cluster* all'interno del «Processo di Oslo», evidenziando l'esigenza che le iniziative del nostro Governo siano assunte sempre in stretta concertazione con i nostri *partner* nell'ambito delle operazioni di pace, si svolgano esse sotto l'egida delle Nazioni Unite, dell'Unione europea ovvero dell'Alleanza Atlantica, rispetto alle quali noi siamo espressione fedele di un concerto internazionale. Sono infatti fermamente convinto che la delicatezza estrema nella quale le operazioni di pace si svolgono richieda il costante rispetto delle esigenze di integrazione reciproca tra i nostri *partner*. Questa forse è la differenza fra la nostra azione di concertazione di un Governo che agirà seguendo questa linea e la vostra concezione di opportunità. Per ragioni analoghe il divieto della produzione e dell'utilizzo delle munizioni *cluster* non può peraltro che trovare compimento in una convenzione che origini dal pieno coinvolgimento dell'intera comunità internazionale.

Sono questi i capisaldi della mozione sulla quale la maggioranza, convinta, voterà a favore. Personalmente esprimo, e lo ricordo ancora, ancora, l'auspicio che si possa pervenire anche in quest'Aula ad un voto dalla forte connotazione *bipartisan*. Sono fiducioso che su questo documento, come avvenne già alla Camera nella scorsa legislatura, si possa registrare un'ampia convergenza di consensi. L'amicizia e la stima che mi legano ai colleghi di minoranza e di maggioranza tutta che l'hanno firmato mi rendono certo che tutti condividano il convincimento che un impegno forte e deciso del nostro Governo anche in questo campo contribuisca a testimoniare la sensibilità del nostro Paese e del nostro Governo, nel campo militare, per un cambiamento etico e morale

a confermare ancora una volta il prestigio di cui il Paese gode nell'ambito della comunità internazionale. Mi auguro che vi sia un voto illuminato.

se non vi è la partecipazione di tutta la comunità internazionale il discorso non può avere successo.

La seduta è ripresa. Colleghi, vi chiedo un attimo di attenzione. Risulta alla Presidenza che è in fase avviata una trattativa tra maggioranza ed opposizione per giungere ad un testo condiviso.

rileggendo insieme le mozioni, a trovare una formulazione che può essere condivisa da tutti, e credo che questo sia un momento importante per il Senato. Ringrazio

nel rispetto degli impegni internazionali nelle operazioni di pace delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza Atlantica, anche in relazione alle esigenze di integrazione reciproca, una decisa

al termine dei nostri lavori, certo di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea, desidero esprimere viva soddisfazione per la tempestività con la quale il Senato della Repubblica ha approfondito e offerto il proprio contributo su una questione tanto importante quale l'utilizzo delle cosiddette bombe a grappolo che, per le loro caratteristiche, possono arrecare danno diretto alla popolazione civile ledendo le norme di un diritto internazionale autenticamente umano. L'appello che il Santo Padre ha rivolto agli uomini di buona volontà del nostro tempo penso sia stato accolto da questo ramo del Parlamento con spirito di autentico servizio per la comunità internazionale tutta. Resta il nostro dovere di dare seguito all'indirizzo che il Senato ha deciso di rivolgere al Governo in tutte le sedi dove siamo chiamati a contribuire in modo concreto e fattivo all'edificazione di un mondo più giusto. *(Applausi